10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale

settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» Sette giorni fa abbiamo reso l'ultimo saluto a un protagonista della nostra storia repubblicana qual è stato il presidente emerito Giorgio Napolitano. In quell'occasione

Non voglio oggi ripetere il mio ricordo, perché suonerebbe meno sentito e spontaneo di quanto è stato nel momento in cui gli abbiamo reso gli abbiamo reso l'ultimo saluto. È però con piacere che saluto il figlio e i familiari che sono anche oggi presenti qui al Senato ed è con estrema emozione che ho accolto la richiesta di ricordarlo anche sette giorni dopo con le parole dei rappresentanti dei Gruppi che desidereranno intervenire in

con Giorgio Napolitano è scomparso uno statista italiano ed europeo di grande autorevolezza. La sua visione politica si fondava sulla storia, sul senso dello Stato, sulla comunanza di destino tra Italia ed Europa. Uomo esigente con se stesso e con gli altri, il suo modo di fare politica era l'esatto contrario di quello così diffuso oggi, che genera sfiducia nei cittadini. Non inseguiva il consenso e la popolarità. La sua innata severità era l'opposto della demagogia. Convinto sostenitore del ruolo primario del Parlamento, sia nazionale che europeo, ha mostrato egli stesso, quale Presidente della Repubblica, che una Repubblica parlamentare non è affatto incompatibile con il governare con tempestività ed efficacia, anche in frangenti drammatici della politica e dell'economia. Durante gli anni della sua Presidenza, l'Italia ha avviato riforme strutturali, anche impopolari, più di quanto sia riuscito, ad esempio, alla Francia, Repubblica presidenziale. Nell'unirmi al cordoglio generale e di quest'Aula per la scomparsa del presidente Napolitano, non posso non ricordare che ho avuto l'onore di collaborare con lui in una fase difficile per il nostro Paese, trovando nella sua persona una guida alta e sempre rispettosa dei rispettivi ruoli. Sono particolarmente vicino ai familiari. In quest'Aula, signor Presidente, noi abbiamo commemorato il 20 giugno la figura del presidente Berlusconi; il 28 giugno abbiamo salutato il presidente Napolitano in occasione dei settant'anni dall'inizio della sua attività parlamentare. Oggi commemoriamo il presidente Napolitano. Ho avuto il privilegio di conoscere da vicino entrambe queste personalità e di cooperare con loro in diversi momenti, a volte problematici. Io credo che sia venuto il momento di ristabilire con pacatezza la verità storica, diradando coltri multiple di nebbie artificiali. Entrambi questi grandi italiani hanno avuto il merito di far superare all'Italia un momento di grande difficoltà politica, finanziaria e di credibilità; entrambi - personaggi profondissimamente diversi - agendo con responsabile senso di cooperazione istituzionale. Non mi riferisco ovviamente alla fase precedente, lo sbocco ultimo delle difficoltà di quel momento, ma mi riferisco alla fase in cui avvenne la transizione dal Governo Berlusconi 2008-2011 al Governo successivo. Questa sarebbe avvenuta, secondo alcuni, contro la volontà dell'allora Presidente del Consiglio. Così dicendo, non solo si dice cosa non vera, fa anche torto non a una, ma a due personalità. Si fa torto al presidente Napolitano, che non ha imposto alcunché a nessuno e che, con la sua autorevolezza e la sua capacità di persuasione, in una situazione in cui l'Italia era profondissimamente spaccata - non contano ora

con gli esigui poteri del Capo dello Stato, è riuscito a creare la cosa più preziosa: un consenso nel Parlamento e nel Paese perché si superassero quelle difficoltà. luogo, non si rende giustizia al presidente Berlusconi con quella tesi secondo la quale sarebbe stato vittima di un complotto, anziché persona che ha saputo mettere in quella circostanza l'interesse del Paese al di sopra dei propri interessi politici e personali. Credo di essere stato un testimone molto prossimo di quelle giornate e il presidente Berlusconi fu protagonista di quella transizione. Ricordo soltanto che il 9 novembre 2011 controfirmò prontamente, senza esitazioni, un decreto di nomina di un senatore a vita - il sottoscritto - che gli venne

a un pranzo, alla presenza dell'onorevole Alfano e del dottor Letta. In quell'occasione mi incoraggiò a superare le difficoltà che ancora sussistevano alla formazione del Governo e - lasciatemi rivelare questo

tutti, tranne uno, e mi citò un Ministro. Ma io fui in grado di rassicurarlo dicendogli che il Capo dello Stato mi aveva già manifestato il suo chiaro indirizzo che io dovessi assumere quel Ministero *ad interim*. Il passaggio delle consegne avvenne con grande cordialità, forse superiore a quella che ventisette mesi dopo caratterizzò un altro passaggio di consegne all'interno peraltro di uno stesso partito. Il 17 novembre, in quest'Aula, presentandomi per la fiducia, dissi di rivolgere infine un pensiero rispettoso e cordiale al presidente, onorevole dottor Silvio Berlusconi, mio predecessore, del quale mi faceva piacere riconoscere l'impegno nel facilitare in quei giorni la mia successione nell'incarico, e salutai il dottor Letta che sedeva nelle tribune. con questo voglio ricordare che forse negli ultimi anni è stato fatto torto a due personalità - ripeto - profondissimamente diverse, a volte contrapposte, ma non contrapposte in quella fase che fu decisiva per ridare all'Italia la propria unità e la propria piena appartenenza alle istituzioni europee.

non è certo il momento oggi per approfondire i lunghi anni del servizio politico e istituzionale di Giorgio Napolitano. Lo hanno fatto molti di noi in questi giorni. La sua vocazione europeista, la scelta atlantica, la ricerca costante del multilateralismo sono stati il cuore pulsante della sua militanza nella sinistra italiana, alla cui trasformazione si è dedicato con passione, così come il suo lavoro ai vertici dello Stato, che ha difeso con decoro e onore. A me preme qui sottolineare un aspetto particolare, ma non secondario della sua vita: l'amore per la politica e il Parlamento. del suo amore per la politica, come il più alto servizio verso il prossimo e verso i più deboli, e della sua dedizione al Parlamento, sede della sovranità popolare. C'è modo e modo di difendere le Assemblee parlamentari: lui lo ha fatto, in Europa e in Italia, con coerenza e chiarezza, con comportamenti concreti, dagli anni della giovinezza (entrò alla Camera a ventott'anni) fino all'ultimo tratto della sua vita.

Da quel giorno, finché le forze glielo hanno consentito, la sua presenza in Commissione è stata costante, attenta, rispettosa di tutti, come nel suo stile. Dalla ribalta internazionale alla quotidianità dell'oscuro lavoro parlamentare, il comportamento di Napolitano non ha mai registrato cali di tensione: tanto era il valore da lui attribuito al Parlamento. La sua curiosità verso i colleghi, soprattutto i più giovani e i più distanti politicamente da lui, hanno spesso alimentato la nostra attenzione, così come i suoi rimbrotti severi e affettuosi, nello stesso tempo, diretti in particolare a chi riteneva più amico. La difesa del Parlamento è coincisa con la difesa della Politica, con la p maiuscola, anche nelle sue prerogative rispetto a invasioni improprie di una magistratura di cui peraltro ha sempre difeso l'autonomia. Non ha indugiato in facili conformismi, anche a costo di sfidare una certa deriva populista da cui, per stile personale e per vocazione politica, non poteva che sentirsi agli antipodi. La strada - sono sue parole - è quella di una dialettica democratica e non quella avventurosa e deviante della contrapposizione tra piazza e Parlamento. E, ancora, il riferimento alla mitologia che si fa della rete: essa fornisce accessi preziosi alla politica, ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace per la formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi e vincolati all'imperativo costituzionale del metodo democratico. l'impegno e la sfida nello stesso tempo ad essere migliori e a trovare le forze per affrontare i pericoli di un tempo perché - come disse sempre in quest'Aula - non possiamo certo evadere, non possiamo scappare, ma siamo chiamati a fare il nostro dovere non come esponenti di una o di un'altra fazione, ma come depositari della volontà popolare. parole monito per tutti noi e credo per le giovani generazioni.

di Giorgio Napolitano. Dire che la sua vita si è intrecciata con l'intera storia della Repubblica non è una iperbole. Quando ci si trova di fronte a una simile biografia è inevitabile il rischio di rendergli un omaggio sincero, ma anche agiografico, mettendo da parte i conflitti, le contraddizioni e anche gli errori che segnano l'esistenza di chiunque come Napolitano abbia inteso la politica in una maniera così totalizzante. Lo è per chi condivideva la sua visione della sinistra che, pur dentro la tradizione comunista in quella generazione e in quel gruppo dirigente che contribuirono a rendere grande il nostro Paese, ne rappresentò per molti versi, se non una rottura, certamente qualcosa in più di una semplice articolazione. Lo è per chi ritiene che la sua idea di Presidenza della Repubblica, segnata da un inedito interventismo, fosse una necessità dovuta alla debolezza estrema della politica di una Repubblica forse mai così fragile come in quel momento. Ma lo è anche per chi nel mondo progressista non condivise - anche io, a volte, fra questi la direzione verso la quale Giorgio Napolitano, da dirigente politico prima del PCI e poi del PDS, pensava fosse giusto indirizzare la sinistra italiana e ha nutrito dubbi sull'interpretazione certamente assai decisionista del ruolo stesso di Capo dello Stato. Personalmente credo che da questo rischio si debba invece provare a rifuggire. Proprio perché la traiettoria politica di Giorgio Napolitano si sovrappone così completamente con la storia della Repubblica, cogliere le domande che lui si è posto e individuare i nodi che ha tentato di sciogliere sono più importanti e più fecondi - io credo - dello schierarsi a favore o contro le risposte che a quegli interrogativi ha dato. Quelle domande e quei problemi irrisolti sono infatti ancora adesso più che mai attuali ed urgenti. Come dirigente del PCI, Napolitano è stato avversario di quella concezione di una certa diversità comunista che, nella cultura politica del partito, era invece predominante; ne vedeva, non senza ragioni, i rischi dell'isolamento politico e di un'idea dell'appartenenza che considerava inefficace. Penso però che non valutasse sufficientemente il rischio opposto, quello di una normalizzazione che avrebbe finito col negare la ragion d'essere stessa di una identità politica. Eppure, il nodo ancora oggi irrisolto della sinistra italiana resta esattamente quello con cui si misurò Giorgio Napolitano. Come incarnare, cioè, le istanze di cambiamento e la visione di un'altra idea del mondo e della politica, senza per questo rinchiudersi in un isolamento autoassolutorio? Come fare politica, cioè, con realismo, senza per questo sacrificare la propria identità? La debolezza della politica, che permise e rese forse inevitabile una centralità del Quirinale fino a quel momento inedita, è ancora evidentemente ben presente, se non ormai del tutto endemica. Il presidente Napolitano ne era consapevole e lo disse severamente al Parlamento - lo ricordiamo tutti - nel discorso che tenne dopo la rielezione. Disse che erano urgenti riforme profonde e, dopo dieci anni, quelle parole hanno ancora una forte attualità. Eppure io credo che si debba provare a ragionare su cosa si intenda per riforme utili a riparare i guasti che denunciò quel giorno Napolitano, senza illudersi, cioè, che scorciatoie salvifiche, imposte magari con un pugno di voti in più, siano quelle giuste. Non sarà sufficiente alcuna riforma senza che la politica smetta di rappresentare un mondo sideralmente distante dalla vita delle persone, per tornare a essere rappresentanza reale di interessi, problemi e questioni reali. Al di là di ogni dissenso, anche quelli più profondi, Giorgio Napolitano da questo punto di vista è stato senz'altro un esempio. Nella sua lunghissima parabola politica nessuno, neppure il critico più aspro, ha mai potuto accusare di essere mosso da un'ambizione personale o di assumere posizioni dettate dal calcolo e dalla convenienza, e men che mai, naturalmente, dall'opportunismo. Non nego certo che, a mio parere, dieci anni fa il presidente Napolitano non colse fino in fondo l'istanza di cambiamento che pure in quel momento animava il Paese. Ne vide solo gli aspetti più populisti e più pericolosi, che pure c'erano, ma non quelli più vitali e democratici, che probabilmente erano invece prevalenti. Così facendo, credo, si perse un'occasione preziosa per rinnovare la nostra democrazia. Ma cito proprio quello che considero un errore per segnalare che, anche quando il dissenso - come in quel caso - è stato profondo, siamo sempre stati consapevoli che a muovere le sue scelte era la limpida convinzione che quello fosse l'interesse del convinzione che quello fosse l'interesse del Paese, non di una parte e nemmeno della sua parte. Così lo voglio ricordare oggi, rivolgendo alla sua famiglia, ai suoi cari alla sua comunità politica le più sentite condoglianze del mio Gruppo parlamentare e dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

ringrazio la presidente Unterberger e i colleghi del Gruppo Per le Autonomie per aver lasciato a me l'onore di ricordare Giorgio Napolitano in Aula, anche a nome del Gruppo. Il presidente Napolitano, infatti, aderì a questo Gruppo quando fece il suo ritorno in Senato, il 14 gennaio 2015, a seguito delle dimissioni da Presidente della Repubblica, e da allora ne ha fatto parte ininterrottamente. Fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito, il Presidente è stato una figura presente e disponibile alle richieste di suggerimenti e confronto da parte di tutti i senatori del Gruppo. La sua presenza è stata sempre e giustamente motivo di grande orgoglio per il Gruppo Per le Autonomie, anche per via dello storico legame che intercorre con i senatori a vita, gli ex Presidenti del Consiglio e i Presidenti emeriti della Repubblica. In questa antica consuetudine, crediamo vi sia la volontà di segnalare al Parlamento come il rispetto delle minoranze costituisca un elemento essenziale per misurare lo stato di salute delle istituzioni. Da Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, definì l'Alto Adige un modello di integrazione pacifica, di convivenza e sviluppo condiviso tra etnie, nazionalità, lingue e tradizioni diverse, che ha dimostrato nei fatti - queste ancora le sue parole - come sia possibile superare ogni livello di conflitto. Passo ora a un ricordo più personale del presidente Napolitano, che risale all'agosto di dieci anni fa. Ricordo ogni attimo di quell'incontro nel suo studio al Quirinale, quando ancora non avevo idea del perché fossi stata convocata. Ricordo di essermi sentita di fronte a un gigante della nostra vita istituzionale e civile. Poi ci fu il momento in cui mi rivelò il motivo di quel colloquio, la sua volontà di nominare i nuovi senatori a vita, e il mio successivo lunghissimo silenzio, quasi prossimo a un mancamento, con tanti pensieri che si accavallavano e che andavano dalla ricerca sulla malattia di Huntington, alla quale ho dedicato la mia vita, ai giovani del mio laboratorio, che stavano costruendo il loro futuro, alla mia famiglia e a questo luogo dove mi trovo oggi a parlare: per me sacro, ma allora sconosciuto. Ricordo le sue parole, quando mi chiese di continuare a essere una scienziata attiva, dentro e fuori il laboratorio, ma contribuendo ai lavori del Senato della Repubblica italiana. Mi fu chiaro che, attraverso la mia nomina e quella di Claudio Abbado, Renzo Piano e Carlo Rubbia, il Presidente volesse richiamare il mondo scientifico e della cultura italiana a contribuire, a sentirsi più partecipe e responsabile del processo democratico parlamentare che conduce alle decisioni pubbliche. Mi fu chiaro che questo per me poteva solo essere un impegno serissimo, che toccava la mia passione più grande, ancora più della scienza: l'impegno civile e la possibilità di contribuire a costruire una società più informata e competente. Nei primi passi nel mondo, a me allora ignoto, della vita parlamentare la vicinanza del presidente Napolitano, fisica in Aula e morale nei momenti in cui ne ho sentito la necessità, è stata fondamentale. Con la sua intelligenza, il senso di responsabilità e la profonda cultura delle istituzioni, mi ha insegnato più di quanto io possa riassumere qui in pochi minuti. Pensare alla fortuna di aver potuto sedere per qualche tempo in Senato accanto a lui e di aver potuto apprendere tanto dal suo esempio e dalla sua viva voce è per me un modo di consolarmi, almeno in parte, della consapevolezza che non sia più fisicamente tra noi. L'eredità morale che il presidente Napolitano ci lascia è nella sua idea della politica quale strumento per il superamento delle iniquità economiche e sociali; nella sua idea delle istituzioni come fondamenta per il perseguimento dell'interesse generale; nella sua idea della Costituzione come promotrice del benessere e della coesione sociale. Rimarrà il ricordo di un Presidente autorevole e rigoroso, ma sempre profondamente umano e capace di interpretare con acutezza i fenomeni della vita politica. Nel concludere, vorrei indirizzare un pensiero affettuoso, da parte mia e del Gruppo per le Autonomie, ai familiari del presidente Napolitano, che onorano oggi quest'Aula assistendo a questa commemorazione. E un pensiero affettuoso anche a tutto il suo *staff*. Da parte mia, resterà sempre forte la memoria della sua vicinanza e della sua disponibilità e sarò sempre grata di aver avuto, da cittadina, il privilegio di essere stata sua compagna di banco negli ultimi anni in Senato.

il presidente Giorgio Napolitano è stato il primo Presidente della Repubblica eletto per due volte ed ha esercitato il suo servizio in un momento molto difficile della storia del Paese, con sei Governi che si sono succeduti. È stato Presidente della Camera in un periodo drammatico, succedendo a Oscar Luigi Scalfaro dopo la sua elezione al Colle. È stato Presidente del Senato e, come fu notato dalla presidente Alberti Casellati appena eletta, fu il primo a ricoprire tutte le tre più alte cariche dello Stato. È stato Ministro dell'interno e credo che la sinistra dovrebbe riflettere su come egli ha esercitato quell'incarico, tra il 1996 e il 1998; erano i tempi in cui vinceva Tony Blair. Legge e ordine erano le parole con le quali la sinistra vinse in Regno Unito; poi non ha più vinto: un motivo ci sarà. è stato tante altre cose. All'interno del Partito Comunista Italiano, è stato un pioniere e un ispiratore, anche quando era in minoranza. Giorgio Napolitano, però, è stato profondamente un uomo delle istituzioni, come lei, signor Presidente, ha ricordato. allora che, anziché fermarsi sui ricordi personali che ciascuno di noi naturalmente porta nel proprio cuore, le commemorazioni servano per ragionare del futuro. Napolitano non è semplicemente un uomo del passato, ma ha ancora qualcosa da dire e da dare per il futuro. Il 29 giugno 2025, quando mi auguro che quest'Assemblea ricorderà il centenario della nascita di Napolitano, mi piacerebbe che il Governo fosse presente nell'individuare alcuni segni concreti della memoria politica che egli lascia a questo Paese. Io ne individuo soltanto tre, signor Presidente, per ragioni di tempo, ma naturalmente saranno altri a farlo più autorevolmente di me nei prossimi anni. Il primo: Giorgio Napolitano è stato uomo dell'Europa anche quando la sua parte politica non credeva all'Europa, ed è rimasto uomo dell'Europa anche quando la maggioranza del Paese iniziava a stancarsi dell'Europa. Si appassionava del futuro dell'Europa forse più di qualsiasi altro argomento. Mi piacerebbe che vi fosse, da qui al biennio che ci separa dal ricordo del suo centenario, un momento nel quale la politica italiana sia all'altezza di quella straordinaria preparazione e visione che il presidente Napolitano aveva sulla necessità per l'Europa di essere non soltanto un luogo di burocrazia e ideologia, ma un luogo di carne viva della politica. Il secondo lo dico sapendo di toccare un tema delicato in quest'Aula e soprattutto per una parte di quest'Assemblea: c'è stato chi, negli anni soprattutto nel 2011, ha pensato che Napolitano esorbitasse dal suo ruolo di Presidente della Repubblica e chi ancora oggi, attaccandosi a una visione formale e direi abbastanza superficiale, continua a fare del Presidente della Repubblica una figura dai contorni Giorgio Napolitano può essere apprezzato o meno nelle scelte che ha fatto, ma si è fedelmente attenuto a poteri costituzionali che la migliore dottrina spiega essere a fisarmonica: non è Napolitano che è andato oltre i suoi poteri; è la Costituzione italiana che oggi prevede per il Presidente della Repubblica poteri e responsabilità allargabili, estensibili e meno ampi sulla base della sensibilità personale o dell'oggettiva situazione politica. Finché non si ha il coraggio di dire che in Italia si può arrivare fino a un semipresidenzialismo di fatto, seguendo la lettura precisa e puntuale della Carta costituzionale, fino all'idea del Presidente del Consiglio come mero arbitro e notaio; finché non abbiamo il coraggio di dire che c'è quest'ampiezza di poteri del Presidente della Repubblica, non si tocca il vero, secondo grande lascito di Napolitano che vorrei restasse in quest'Aula: Napolitano era un uomo che voleva le riforme costituzionali perché, pur convinto che la nostra fosse la Costituzione più bella del mondo, ne vedeva i limiti. Non avere il coraggio di dire che toccare questo tema significa toccare un grande punto aperto della politica italiana significa non essere seri con noi stessi. Se volessimo davvero essere intellettualmente onesti con la memoria di Napolitano, questo - che pure in alcuni casi ha visto anche profonde discussioni con lui, com'era giusto e doveroso che fosse - è un tema, il tema. La figura del Capo dello Stato non può essere utilizzabile per attaccare semplicemente per ragioni personali o politiche; è una figura i cui confini i cui contorni richiedono una precisazione costituzionale. Terzo e ultimo punto: Napolitano era un uomo che credeva nella giustizia giusta e che ha subìto negli ultimi anni della sua vita - o meglio, più correttamente, negli ultimi anni del suo magistero al Quirinale - una drammatica vicenda personale.

dalla Corte di cassazione, su cui il Presidente della Repubblica fu chiamato a rispondere, ancorché nella sede del Quirinale. Io sono stato testimone della sofferenza personale e familiare che quella vicenda ha prodotto. Naturalmente, nessuno di noi ha dubbi, anche alla luce dell'esito giudiziario della vicenda, ma bisogna avere il coraggio di dire che, quando si sceglie il giustizialismo contro le garanzie della Costituzione e del mondo della giustizia, si produce una sofferenza alle persone e alle loro famiglie che troppo spesso viene sottaciuta

di prendere atto che, di fronte a questa figura così rilevante delle istituzioni, l'ultima cosa che si può fare è darne un giudizio superficiale o banale, perché, se c'era una cosa che Napolitano odiava più di qualsiasi altra, era la sciatteria, la mancanza di attenzione nello studio e nella capacità di approfondire. Quando il presidente Napolitano ti chiamava a confrontarsi su un punto, sapevi che avevi a che fare con un uomo che entrava nel merito dei problemi e ti sfidava al livello più alto. Siamo all'altezza di questo ricordo, non limitiamoci ciascuno a fare il proprio compitino, ricordando in un'occasione o in un'altra. Il presidente Napolitano è stato un gigante di queste istituzioni; dedichiamoli pure tutte le aule e i luoghi istituzionali che vogliamo, ma sappiamo che il suo è un messaggio di sfida alla politica, perché egli era un uomo che amava la politica almeno quanto amava la vita. Senatore Renzi, il Governo per fortuna era rappresentato quasi al completo sette giorni fa. È corretto da parte mia ricordarlo.

combattuto buone battaglie, sostenuto cause sbagliate e cercato via via di correggere errori e di esplorare strade nuove. Sono parole di Giorgio Napolitano citate da suo figlio, secondo cui la vita politica di tanti protagonisti conosce trasformazioni, errori e innovazioni. In questa sede, non devo ricordare la intensa biografia politica di Giorgio Napolitano che poi nel suo schieramento, con i miglioristi, con una componente riformista, cercò di innovarne il percorso, tuttavia egli stesso ricordava in quest'autobiografia storie lontane. Oggi siamo qui per una commemorazione; questo non è un convegno, non dobbiamo rianimare polemiche e riaprire ferite su storie della vita politica recente che hanno fatto e faranno discutere, che hanno prodotto libri, polemiche, analisi interne e internazionali. Ritengo però che il fatto di credere alla lotta politica - un'affermazione che condivido - nobiliti chi partecipa in maniera attiva e convinta. Lei ricorderà, signor presidente La Russa, che all'inizio della scorsa legislatura il presidente Napolitano presiedette per ragioni anagrafiche, e non solo per il prestigio della sua storia, la prima seduta del Senato. Io gli chiesi, con fare un po' sfrontato, se potevamo fare una fotografia

presidente Napolitano c'è stato anche scontro politico, ma non voglio parlare di quello recente. Ad esempio, quando ero un giovane parlamentare, nella legge Turco-Napolitano c'era scritto che gli immigrati extracomunitari potevano votare alle elezioni amministrative. Ciò non era conforme alla Costituzione, ci fu uno scontro - io ero giovane, lui era già autorevole

Ci fu uno scontro morale, direi etico, su princìpi diversi, proprio perché Napolitano interpretava una sua storia, una sua cultura e una sua parte politica. Le altre vicende le tralascio. Il presidente Monti ha fatto una sua ricostruzione. Concordo con Gianni Letta, che ha detto il presidente Napolitano non esercitò un ruolo meramente notarile. Se l'ha detto Gianni Letta, moderato tra i moderati, si può dire. Io, che ero Capogruppo in quegli anni e che con Napolitano ho parlato di tutto della Corte costituzionale, dei Governi, dell'andamento dei lavori parlamentari - non mi sono meravigliato, perché ritengo che un ruolo non notarile il Presidente della Repubblica lo eserciti. Parlammo anche di persone, di nomi e di situazioni con la riservatezza che mantengo ancora oggi, perché ognuno esercita i ruoli secondo una certa etica. Poi le cose sono andate come sono andate, dopodiché, dallo scontro su alcuni temi

l'improvvisazione non paga mai, cari colleghi, e che si impara sempre qualcosa nel confronto del Parlamento e della democrazia anche dal proprio avversario, che può rimanere distinto e distante, ma con il quale in questo luogo si può combattere, discutere e capirsi. Con questo spirito non servile, ma sincero, il Gruppo Forza Italia si unisce al ricordo del presidente Napolitano. Presidente, senatrici e senatori, quando un feretro sfila perché un cuore ha cessato di battere, niente vale di più dell'umana espressione di cordoglio e di vicinanza ai familiari. Questo è stato detto e questa è la prima cosa da dire. Oggi siamo chiamati ad esprimere una riflessione su una delle figure politiche più importanti del secolo scorso. Noi crediamo che la forma migliore per portare stima e ossequio sia quella di potersi esprimere nella maniera più rispettosa possibile, ma anche nella maniera più sincera possibile. Qualcuno poc'anzi in Aula, nel suo ricordo, ha evocato la dote della schiettezza, che fu la costante del suo portato politico e umano. Ebbene, è nel nome di quella stessa schiettezza che il MoVimento 5 Stelle oggi non si nasconderà dietro il velo dell'ipocrisia con mutate valutazioni o, peggio, incoerenti rispetto a quello che è stato un giudizio politicamente negativo che abbiamo sempre espresso su Giorgio Napolitano con lealtà e con trasparenza. Questo perché, a distanza di anni ormai dal termine del suo lungo mandato, resta ancora forte e diffuso il nostro ricordo delle sue costanti, talvolta pervicaci, refrattarietà e riluttanza a tutto ciò che poteva ricondursi alla parola «cambiamento». Eppure, egli accettò di traghettare l'Italia attraverso anni di forti istanze di cambiamento. Erano voci di una fase storica di grande riflessione civile; voci, però, che lui non seppe o non volle ascoltare. Le risposte deludenti della politica di allora di fronte ai tanti scandali pubblici, alle deviazioni di apparati dello Stato e agli intrighi di potere non lo trattennero

ma nemmeno la conclamata incapacità della politica di quegli anni di autoemendarsi e di autocurarsi dal cancro delle tangenti, dalla corruttela e dall'omertà lo indussero ad aprirsi o ad aprire una fase e un processo di revisione critica verso una classe politica e verso una fase politica tutti vedevano ormai prossima al collasso, e così fu qualche anno dopo, con il ciclone di Mani pulite. Egli accettò di restare al centro della scena politica in una delle crisi più tragiche - lo avete detto della storia repubblicana, ma lo fece interpretando quelle forti spinte civili e sociali come meri pericoli per la stabilità dello Stato e, nel suo sforzo e, nel suo sforzo di difendere la Costituzione, finì per travalicarne i perimetri, smettendo piano piano i panni del rappresentante di Stato per divenire egli stesso Stato. Furono gli anni in cui «The New York Times» lo battezzò re Giorgio. È questo È questo il nostro giudizio politico di un uomo colto, attento, abile e capace, ma che volle farsi re per difendere la Repubblica da se stessa. Di lui, tuttavia, resta l'amore per la sua Patria per la Nazione e tanto basta perché il MoVimento 5 Stelle renda oggi onore al senatore Giorgio Napolitano. Signor Presidente, oggi commemoriamo il presidente emerito Giorgio Napolitano, una figura di grande rilevanza nella storia politica italiana. Pur provenendo da diverse appartenenze politiche, riconosciamo tutti l'importanza del suo contributo al nostro Paese e alla politica italiana nel suo complesso. Giorgio Napolitano è stato un uomo che ha dedicato la sua vita intera alla politica, con un amore profondo per la politica di partito, quella fatta di sezioni e di militanza, concetti che oggi sembrano essere in declino. Questo è un aspetto fondamentale della sua eredità, che vorrei sottolineare oggi: la politica di partito, la politica di parte, la politica di sezione e di militanza è certamente ciò che ha caratterizzato Giorgio Napolitano nella sua lunga vita ed è una politica che può ancora oggi essere un veicolo per il cambiamento positivo, se abbracciata con un profondo senso di responsabilità e dedizione al bene comune. Il radicamento nelle comunità locali, la capacità di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo dato alla formazione di nuove generazioni di politici e *leader*, in un'epoca in cui la politica è accusata di essere più distante dai cittadini, nonostante i nuovi mezzi di comunicazione ci illudano in qualche modo di comunicare più velocemente con il nostro elettorato, le tradizioni politiche di lungo corso e la militanza nei territori rappresentano ancora il vero modo per mantenere un legame forte con la vita quotidiana del Paese e dei cittadini. Dobbiamo recuperare quell'amore per la politica basata sul servizio pubblico, sull'ascolto delle esigenze dei cittadini e sulla ricerca di soluzioni che possano migliorare le loro vite. È importante ricordare allo stesso tempo che proprio il suo essere di parte ha fatto sì che i suoi incarichi istituzionali non siano stati privi di controversie. Una delle situazioni più discusse è stata senz'altro la sua reazione alla crisi politica del 2011, a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e l'incarico conferito all'ex commissario europeo, oggi senatore a vita Mario Monti, per formare un governo tecnico. Non possiamo ignorare il fatto che quella situazione abbia sollevato interrogativi sulla sua interpretazione del ruolo istituzionale. Lo stesso vale per l'aperto sostegno all'intervento militare in Libia, sempre nel 2011, di fianco agli alleati occidentali o la gestione della dolorosa vicenda umana di Eluana Englaro, con la lettera inviata all'allora presidente del Consiglio e poi con il rifiuto di firmare il decreto del Governo, causando uno scontro istituzionale forse senza precedenti. Ancor prima - e noi leghisti ce lo ricordiamo bene - vi fu la perquisizione nella sede di via Bellerio il 18 settembre 1996 (tre giorni dopo la grande manifestazione della Lega sul Po), Lega sul Po), che portò al ferimento del nostro Roberto Maroni e di alcuni dirigenti, mentre Napolitano ricopriva l'incarico di ministro dell'interno. L'interpretazione interventista e politica del ruolo presidenziale ha suscitato dibattiti accesi e critiche; la discussione su come interpretare correttamente il ruolo della Presidenza della Repubblica è parte integrante del dibattito e costituisce un aspetto importante della sua eredità. Questi ragionamenti utili per mantenere in salute lo stato della nostra democrazia non vogliono in alcun modo negare la dedizione del presidente Napolitano nei confronti della causa pubblica e il suo contributo alla storia del nostro Paese, che rimarranno un segno importante nel panorama politico italiano. Un'ultima riflessione, prima di concludere: senza dubbio, la vita politica sempre dichiaratamente di parte di Giorgio Napolitano è stata caratterizzata da una serie di fasi e di sviluppi, tra i quali troviamo il suo sostegno da giovane alla repressione sovietica in Ungheria del 1956, seguito dal suo atto di pentimento e omaggio alla resistenza ungherese durante la sua presidenza. Questo percorso di evoluzione delle idee è emblematico della complessità della politica e della natura stessa della crescita e della maturazione di un individuo. È innegabile che per ogni politico decisioni o posizioni passate, alla luce di nuove esperienze e riflessioni, possano apparire controverse e sbagliate. Tuttavia, è altrettanto importante riconoscere la capacità di un *leader* di ammettere tali errori ed impegnarsi per il cambiamento positivo. Nel caso di Napolitano, il suo atto di omaggiare la resistenza ungherese è stato un gesto significativo di pentimento e riconciliazione con la storia. Questo ci ricorda che nessuno è immune dagli errori e che l'importante è la capacità di imparare da essi e di crescere come individui e *leader*. Nel contesto della politica, in cui le decisioni possono avere conseguenze significative per intere Nazioni, la maturazione delle idee è un segno di saggezza e di integrità. Perciò, invece di rincorrere gli scheletri nell'armadio di chiunque (tendenza quanto mai attuale e preoccupante), è importante valutare il modo in cui un individuo, soprattutto impegnato nella politica, ha sviluppato le sue opinioni in risposta alle sfide e alle esperienze che ha affrontato. Questo processo di crescita e di maturazione è è essenziale per la politica e per il miglioramento continuo delle decisioni che influenzano la vita di molti. Concludo il discorso esprimendo, a nome di tutto il Gruppo Lega del Senato, le più sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio Napolitano e a tutta la sua famiglia politica. Che riposi in pace.

settantasette anni di storia: la Repubblica inizialmente in fasce, che muoveva i primi passi; la Repubblica delle grandi trasformazioni; la Repubblica del *boom* industriale; la Repubblica delle grandi crisi e delle grandi rinascite. Giorgio Napolitano ha accompagnato la Repubblica in un'Europa che inizialmente non c'era, che poi è diventata stella polare Giorgio Napolitano, come ha ricordato il figlio Giulio - che il Gruppo Partito Democratico saluta e abbraccia con tutta la famiglia la famiglia - entrò durante la guerra nel Partito Comunista come tanti giovani di allora; non era attratto certo dall'Unione Sovietica, ma quel partito gli era sembrato l'organizzazione più adeguata per combattere il fascismo. Sì, signor Presidente, perché l'impegno politico e civico di Giorgio Napolitano nacque in quel momento storico e poi quel partito, quello togliattiano, che dopo il 1944 scopriva il popolo, gli era sembrato nella realtà napoletana di allora il più attrezzato per rimettere in piedi la democrazia italiana. In quel contesto, colleghi, maturò quel patrimonio culturale del suo riformismo, quella competenza che si deve unire alla capacità di cambiare in meglio l'esistente, che si legò sempre all'ideale europeo che caratterizzò di fatto l'impegno di Giorgio Napolitano in tutto il suo percorso politico: il sentirmi europeo, il rapporto con la realtà dell'Europa e con il progetto dell'integrazione e unità europea - scriveva nel 2016 ha rappresentato uno snodo essenziale della mia esperienza nel suo graduale evolversi e nel suo profondo rinnovarsi. Grazie a lui e a tanti altri quel partito, il Partito Comunista Italiano, prese la strada per iniziare il percorso che lo portò ad entrare nella famiglia del socialismo europeo. Primo Presidente della Repubblica a venire dalla tradizione comunista, è stato essenzialmente uomo delle istituzioni. Prima da uomo di partito, capace di posizioni diverse rispetto alla cosiddetta linea, ma sempre senza alzare la voce o minacciare scissioni, perché si può stare in una comunità politica anche in minoranza, anche senza condividere la linea della maggioranza, ma combattendo per ideali che nel lungo termine e indicano la strada più giusta. Poi parlamentare, Presidente della Camera, Ministro e Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, signor Presidente, è stato un uomo di Stato, tra i primi a comprendere le difficoltà, a individuare le crepe nel nostro sistema democratico, consapevole della necessità di riforme strutturali del nostro sistema politico. Le sue scelte hanno sempre avuto come stella polare la difesa della nostra Costituzione e la tenuta del tessuto democratico anche nei momenti più difficili. più difficili. Signor Presidente, tra le tantissime proposte di legge, molte delle quali trasformatesi in legge, ne abbiamo ritrovate alcune che ci piace ricordare oggi, nel giorno della sua commemorazione: una sua decretazione d'urgenza, che dovrebbe farci riflettere; una sulla riforma dell'università e alcune parole sul diritto allo studio; quella sulla contabilità generale dello Stato, che sta particolarmente a cuore a me, perché l'ho utilizzata nella riforma del bilancio che per cento del Parlamento approvammo nel 2016. Nel lontano 1983, signor Presidente, Giorgio Napolitano sulla decretazione d'urgenza diceva che la materia aveva perso carattere di straordinarietà ed era divenuta un modo normale di legiferazione, svuotando sostanzialmente il bicameralismo. Lo diceva quarant'anni fa: non avrebbe mai immaginato che un giorno la prassi ci avrebbe portato ad una sorta di monocameralismo alternato, ma è la condizione nella quale siamo.

quarant'anni fa. In tema di bilancio pubblico, con una proposta di legge del 1983, sottolineava l'importanza della legge finanziaria quale strumento finalizzato a porre un freno alla legislazione di spesa, all'epoca già frantumata frantumata e fuori controllo. Sono tanti gli insegnamenti che il presidente Napolitano ci ha lasciato, ma quello che offriamo alla riflessione di tutti i Gruppi parlamentari che oggi lo hanno commemorato è

In quel passaggio, non meno imperdonabile per la classe politica fu il fatto di non essere riuscita a fare un salto di qualità, per infrangere il tabù di un bicameralismo che segnava metteva in evidenza le proprie difficoltà e che di fatto era superato da una prassi che oggi tocchiamo con mano, ma mai, mai, mai, in nessun modo, il presidente della Repubblica emerito Napolitano ha messo in discussione la figura del Presidente della Repubblica come garante dell'unità costituzionale. Noi speriamo che questo insegnamento ci possa illuminare in questo confronto che abbiamo di fronte. Concludo semplicemente ricordando all'Assemblea che nel 2011 a Rimini, davanti a una platea di giovani, in occasione del 150° anniversario della nascita dello Stato unitario, spiegò il filo ispiratore di quelle celebrazioni individuandolo nell'impegno a trasmettere piena coscienza di quello che l'Italia e gli italiani hanno mostrato di essere in periodi cruciali del loro passato e delle grandi riserve di risorse umane e morali, di intelligenza e di lavoro. Con lui, signor Presidente,

scusandomi se lo riceverò con qualche minuto di ritardo, appena concludiamo questa fase dei lavori.

una figura così importante, che ha segnato sicuramente la storia della nostra Nazione, va ben al di là della parte politica nella quale ha militato. La valutazione storica verrà fatta in sede storica, per l'appunto, perché una personalità che ha segnato così profondamente la storia della nostra Repubblica è in quella sede che troverà le sue valutazioni e i giudizi, per comprendere che cosa il suo lascito significherà per la nostra Nazione, oggi e nel futuro. In questa sede, credo che sia giusto ricordare quanto sicuramente ci accomuna e quanto la sua figura possa ispirare chiunque, di qualunque parte politica. Il suo profondo senso delle istituzioni l'ha espresso nel suo lunghissimo impegno politico, impegno politico, cui ha dedicato oltre settant'anni, ai livelli più alti, dalla sua prima elezione alla Camera, che lei, presidente presidente La Russa, volle ricordare in una giornata, il 28 giugno, il giorno prima del novantesimo compleanno del nostro collega oggi scomparso, e tre giorni dopo i settant'anni anni dalla sua prima elezione. L'impegno che ebbe fin dalla sua prima legislatura, la passione e l'attenzione per i lavori parlamentari non lo hanno mai abbandonato durante tutto il suo altissimo altissimo *cursus honorum*. Anche da Presidente della Repubblica seguiva con estrema accuratezza ogni passo dei lavori parlamentari. Ricordo che ero relatore di un'importante provvedimento e le volte che mi era capitato di interloquire con il presidente Napolitano mi accorgevo che conosceva esattamente le posizioni, le proposte e i dubbi di ogni singolo membro della Commissione che si stava occupando occupando di quel provvedimento, senza bisogno di appunti o di altri strumenti per ricordarseli. Un Un atteggiamento tanto coscienzioso, che ha segnato, dandogli una forte impronta personale, tutte le cariche che ha avuto, è stata probabilmente una delle caratteristiche principali del suo impegno politico. Deputato per molti anni, ha ricoperto incarichi importantissimi all'interno del suo partito; Presidente della Camera in un periodo molto difficile e discusso; Presidente della Repubblica, il primo a essere eletto per due volte alla massima carica della Repubblica; e anche, com'è stato ricordato, Presidente del Senato, sia pure provvisorio, nella prima seduta della scorsa legislatura,

cito alcuni elementi che credo ci possano davvero accomunare tutti. Parlando di Europa, ricordò l'importanza delle conquiste che ci sono state negli ultimi decenni e in quelli seguiti alla guerra, con particolare

la conquista della pace: e abbiamo ben visto quanto fossero appropriate queste parole l'anno scorso, quando purtroppo è iniziata una guerra proprio nel territorio europeo. In un passaggio successivo disse che occorre scongiurare la violenza, in tutte le sue motivazioni e in tutte le sue forme. Anche questa parte va messa in relazione con il senso delle istituzioni, che non può che essere rispetto per le istituzioni:

la parte cui appartiene la figura contestata: sarebbero state inaccettabili manifestazioni violente contro il presidente Napolitano; sono inaccettabili le manifestazioni violente che abbiamo visto oggi nei confronti del presidente Meloni a Torino. chiuse la parte principale del suo intervento raccomandando la necessità di rendere più partecipata ed efficiente, attraverso tutti i canali di riforma percorribili, la nostra democrazia nel solco della Costituzione repubblicana. Riconoscendosi in queste parole, il Gruppo Fratelli d'Italia rivolge un pensiero particolare ai familiari del presidente Napolitano qui presenti e a coloro che sono stati particolarmente vicino a lui nell'impegno politico in questo momento di ricordo. finestra"). Prima di passare alla discussione dalla sede redigente dei disegni di legge che concernono

nuova finestra"). Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che nella seduta del 3 ottobre 2023 ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: nella Regione Emilia-Romagna: Alberto Balboni, Michele Barcaiuolo, Lucia Borgonzoni, Pier Ferdinando Casini, Marco Croatti, Graziano Delrio, Marta Farolfi, Silvia Fregolent, Marco Lisei, Daniele Manca, Elena Murelli, Vincenza Rando, Domenica Spinelli e Sandra Zampa.

Ilrelatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. giunge all'esame dell'Assemblea il testo unificato formulato dalla 7a Commissione permanente all'esito dell'esame in sede redigente concluso il 26 luglio scorso. Il testo in esame risulta dalla congiunzione del disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo, con il disegno di legge n. 533, a prima firma del senatore Menia, e con il disegno di legge n. 548 di iniziativa del senatore Gasparri. Il disegno di legge, composto di un unico articolo, apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2004 che ha istituito il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Con una prima modificazione si prevede l'indizione annuale, in occasione del giorno del ricordo, di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in un capoluogo di Regione differente ogni anno. La seconda novella alla legge n. 92 del 2004 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni. Con un'ulteriore integrazione alla legge n. 92 del 2004 è concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ai seguenti beneficiari nella misura di 75.000 euro annui per ciascun soggetto: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale Centro di raccolta profughi l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Infine viene modificato l'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 al fine di prevedere che la domanda per la concessione dell'insegna metallica riconosciuta a titolo onorifico ai congiunti dei soggetti infoibati, in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, possa essere presentata anche dal sindaco del Comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi. Questo per quanto riguarda gli aspetti puramente tecnici. Dal punto di vista politico, avviandomi alla conclusione, signor Presidente, devo ringraziare i miei colleghi della 7a commissione perché il testo finale licenziato è il risultato e l'espressione di una convergenza fra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che la tragedia delle foibe è stata un abisso che ha inghiottito nel suo errore migliaia di italiani vittime della furia ideologica comunista di Tito, che ha travolto e cancellato ogni senso di umanità, la centralità della persona e dei valori di libertà e democrazia e ha costretto centinaia di migliaia di nostri connazionali a esodare dalle terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra: una tragedia e una verità storica per troppo tempo dimenticata, se non ridimensionata o volutamente e vergognosamente oscurata. che la guerra è purtroppo tornata a insanguinare pezzi d'Europa è fondamentale ribadire che la libertà va sempre di pari passo con la verità e che il rispetto della vita di ogni essere umano e dello stato di diritto sono il nostro faro e l'unico baluardo contro ogni forma di barbarie, totalitarismo e violenza.

poi ne portano in sé il ricordo in maniera viva molto più che con lo studio astratto. Potenziare queste iniziative meritorio, soprattutto se lo si fa con delle opere d'arte che coinvolgono le università e che faranno esporre nei Capoluoghi di Regione per un anno queste iniziative degli studenti di architettura e di ingegneria che testimonieranno con la loro fantasia e con il loro valore un nuovo modo di celebrare

modo al Ministero dell'istruzione e del merito di poter organizzare dei viaggi più omogenei e potenziati in tutto il fronte orientale.

in un concetto assolutamente psicopatologico per cui solo le verità belle di una certa parte politica vanno raccontate e le brutte vanno rimosse sempre. Questa ingiustizia storica ce la siamo portata dietro per decenni, aumentando ancora di più il dolore dei sopravvissuti, delle persone care, di chi è stato obbligato ad allontanarsi col cuore spezzato dalla propria terra per una furia comunista, con l'orco Tito.

pulite, aggiungendo dolore a dolore, amarezza ad amarezza, solitudine a solitudine, anche se poi queste persone sopravvissute, piene di dignità, hanno reagito con coraggio, con misura e con onestà, ma il dolore di chi è morto, è stato ucciso, è stato segregato, torturato, abusato non può essere rimosso né assolto in alcun luogo. I luoghi emblematici li ha nominati il relatore: Basovizza, il Museo centrale, i luoghi dell'orrore, piccoli *lager* grandi nel dolore. Io credo che questo provvedimento non restituirà nulla a chi non c'è più, ma

quasi impressa nel DNA, nella genetica di chi sopravvive o di chi sopravvive a chi è sopravvissuto, cioè alle future generazioni. Però a qualcosa serve: a che non si ripeta più e soprattutto serva a portare democrazia e la democrazia è prima di tutto verità storica. Questo finanziamento, che permetterà viaggi,

lo dico senza piaggeria - a parte il relatore e chi, con

il senso di quello che è accaduto, e che ancora sta accadendo finché qualcuno dirà ancora l'ultima bugia o un'ultima rimozione ipocrita, come il senatore Menia, ha fatto del dolore che rappresenta e che prova una poesia, una musica difficile

hanno vissuto e non vivono in quel periodo, ma che hanno sempre la sensazione di poter fare in futuro qualcosa in più. Io sono felice di parlare con una voce stonata, rispetto alla consapevolezza di tanti altri, di questo provvedimento e di questi fatti, di questi accadimenti.

e delle stelle taccia per un istante, perché l'orrore provocato alle genti, alla collettività, sia contro natura e quindi anche la natura taccia per un secondo. Ecco, io credo che oggi non dobbiamo tacere nemmeno un secondo, ma essere indignati per chi ha parlato troppo poco,

che questa volta, ancora una volta, il Senato, o almeno una parte di esso (anche se spero di no) ha parlato, in maniera consapevole e dolorosa, il lessico difficile ma miracoloso e meraviglioso della democrazia, anche se si interviene troppo tempo dopo. Questo comunque non diminuisce il valore del provvedimento che,

Per evitare fraintendimenti o equivoci, in buona o in cattiva fede, vorrei chiarire subito alcuni punti essenziali. Noi ci riconosciamo nelle parole pronunciate alcuni mesi fa dal presidente Mattarella, quando sottolineò la finalità del Giorno del ricordo, così come indicata nella stessa legge istitutiva: «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». «Un carico di sofferenza, di dolore e di sangue - aggiunse il Presidente - per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e, in certi casi, persino negato». L'ho detto prima e lo ribadisco: mi riconosco e ci riconosciamo pienamente in queste parole. Peraltro, come ho già avuto modo di dire in quest'Aula, penso di poter dire che noi, differentemente da altri, abbiamo fatto da tempo fino in fondo i conti con la nostra storia e quello che contestiamo non sono certamente i fatti, ma una certa interpretazione dei fatti e soprattutto il loro utilizzo storico. La nostra scelta di astenerci non è motivata né da reticenze e nemmeno da ambiguità sul giudizio storico nettissimo che diamo sulle uccisioni, sull'esodo e sulla pluridecennale rimozione di quella tragedia, tragedia, che credo vada inquadrata dentro la complessa vicenda del nostro confine orientale. La storia non è uno spezzatino, non se ne scelgono alcune parti tralasciandone altre: l'italianizzazione forzata, l'invasione della Jugoslavia, i massacri nazifascisti sono parte di quella storia e non possono essere espunti, ma non voglio in alcun modo che questa rivendicazione di onestà storica possa passare per giustificazionismo, anche se non manca certamente chi l'ha usata tendenziosamente. Le catene di violenze e di soprusi precedenti - che sono reali - non possono essere dimenticate, ma neppure utilizzate per giustificare quello che non è in alcun modo evidentemente giustificabile; quindi nessuna reticenza sul giudizio storico. I nostri dubbi riguardano piuttosto l'uso della memoria, in questo come in altri frangenti. Tutti esaltiamo spesso il valore della memoria e io penso sia giusto e necessario farlo. Sarebbe però ora di fare un passo avanti e dire chiaramente, Presidente, che della memoria si può fare buon uso, ma se ne può fare anche uno cattivo. La politica italiana, larga parte della politica italiana è stata negli ultimi anni maestra nel fare il peggior uso possibile della memoria e della storia. Si fa cattivo uso della memoria quando la si usa come un oggetto contundente da adoperare nella contesa politica del presente. Si fa cattivo uso della storia quando la si maneggia non per elaborare e superare lacerazioni, ma per riprodurle all'infinito. Si fa cattivo uso della memoria storica quando la si sfrutta come espediente che assolve dall'obbligo di affrontare la battaglia politica nel presente, appellandosi in questo modo al solo richiamo identitario. Si fa un cattivo, anzi un pessimo uso della storia soprattutto quando si cerca di usare capziosamente singole vicende per insinuare l'idea che nell'immane tragedia del Novecento non ci fossero una parte giusta e una sbagliata. Dunque, il buon uso della memoria non è un esercizio facile. Richiede lucidità, misura e profonda onestà. Bisogna saper prendere in considerazione l'intero quadro complessivo, fuggendo la tentazione di esaltare solo gli aspetti più utili per la propaganda di parte, ma allo stesso tempo rifiutando alla radice ogni giustificazionismo e ogni negazionismo. Bisogna cioè avere il coraggio di ammettere verità che ci feriscono senza dimenticare che, nella più atroce guerra che il mondo abbia mai conosciuto, non si fronteggiavano soggetti equivalenti. Ritengo necessaria questa premessa, perché temo che la proposta di cui oggi discutiamo possa pendere dal lato di un cattivo uso della memoria, non per pregiudizio, ma perché nella proposta di legge non si fa proprio menzione, per esempio, di quelle complesse vicende del confine orientale che invece figuravano nella legge istitutiva del Giorno del ricordo. credo che una cosa sia non adoperare la memoria a fini giustificazionisti, altra evidentemente è espungere oppure cancellare intere e fondamentali parti della storia. il finanziamento per la ricerca storica è indirizzato solo per le associazioni degli esuli, escludendo senza alcun motivo ragionevole gli istituti di ricerca, le associazioni e le fondazioni che, da anni e con gran merito, si occupano delle vicende del confine orientale. orientale. È una scelta davvero inspiegabile se l'obiettivo è quello di restituire al Paese e alle giovani generazioni una memoria storica priva di rimozioni, ma lucida e completa. Allo stesso modo la delega solo alle associazioni degli esuli dei Viaggi del ricordo finirebbe - io credo - per cancellare aspetti di quella vicenda storica che sono invece fondamentali; per esempio, la costituzione delle Repubbliche libere partigiane, tra cui una, quella della Carnia, fu la prima - pensate voi - a deliberare il diritto di voto per le donne nel nostro Paese. Se della storia e della memoria vogliamo fare buon uso, dobbiamo essere capaci tutti di accantonare l'interesse di parte e dobbiamo essere capaci di abbandonare la strumentalizzazione ai fini della propaganda. Le scelte cui ho fatto invece riferimento, senza nulla togliere, a mio parere, all'importanza del ricordo della tragedia delle Foibe e dell'esodo, non vanno in questa direzione; per tale ragione ci asterremo Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, tutte le iniziative di approfondimento di circostanze storiche e di ricordo delle sofferenze patite da esseri umani senza colpa sono fonte di crescita e di arricchimento culturale per le nuove generazioni; sono quindi da sostenere senza discussione. Capisco le considerazioni fatte prima di me dal senatore De Cristofaro e, in qualche misura, colgo anche le criticità Nulla infatti come il confine orientale e le vicende degli anni a cavallo della guerra e nell'immediato Dopoguerra, sono rappresentative di quali tragedie possa provocare la belva umana, come la chiamava Guccini, quando è rappresentata da diverse parti, tutte altrettanto belve che spesso fanno a gara a chi lo è di più. Io ho avuto la ventura di sposare una donna di origine giuliana che, per parte di madre, è di famiglia profuga dell'Istria, e quindi ho avuto la fortuna di poter approfondire direttamente da testimonianze viventi quello che è accaduto

c'erano i cattivi, che erano gli altri, e i buoni, che eravamo noi. Scoprire poi che non è andata proprio così, che ci sono tanti buoni e tanti cattivi di diverse parti, consente però di avere la mente più aperta e più ampia. Sono convinto che anche questa iniziativa possa servire ad aprire la mente dei nostri concittadini del futuro. Nel 1988 insegnavo in una scuola media e organizzai una gita scolastica a Trieste. Andammo a visitare la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza, perché ritenevamo corretto fare questo. Eravamo nel 1988, trentacinque anni fa, molto prima che la Foiba di Basovizza venisse resa accessibile Ricordo che quella fu un'esperienza straordinaria per i miei studenti di allora, che sono oggi quasi cinquantenni. Chiudo nel dare un segno di speranza. Nelle mie esplorazioni della costa dalmata mi è capitato di arrivare a Sansego, un'isola che si trova a sud di Lussino, chiamata il vigneto galleggiante, perché è circa un chilometro quadrato di vigne sopraelevato rispetto al mare Adriatico. Ebbene, in cima a questo pianoro, nel punto più alto, c'è un cimitero, dove ci sono diverse tombe scavate di fresco, con con lapidi di sepolti di lingua italiana, che erano gli abitanti di quella zona che sono andati via da lì, hanno fatto più o meno fortuna, si sono trovati in condizioni all'inizio sicuramente molto difficili, però poi, rimboccandosi le maniche, hanno contribuito contribuito a costruire comunità in giro per il mondo, anche nella mia città, ed infine tornano o si fanno riportare per essere seppelliti in questo luogo con vista sul mare, che ricorda quello che hanno visto tutte le generazioni passate passate delle loro famiglie. Credo che questo sia un segnale che ci dice che, qualsiasi cosa succeda, la si può superare con la buona volontà, con la voglia di lavorare e con la voglia di approfondire culturalmente e come si deve le vicende storiche.

italiana, un massacro iniziato nel 1943 e andato avanti per diversi anni. Proprio mentre il Paese, la maggior parte degli italiani, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, provava a ripartire e a ritornare faticosamente e gradualmente alla normalità, un destino avverso colpiva invece gli italiani nelle terre occupate dalle truppe jugoslave. Queste Queste persone, anziché tornare alla normalità, hanno vissuto una situazione di profonda costernazione, fatta di torture, di carcere, di epurazioni, di morte. Furono coinvolti bambini, donne, giovani e anziani, famiglie della Venezia Giulia, ma anche della Dalmazia, che dovettero sperimentare la disumanità dei totalitarismi del '900. Quella delle foibe è stata una tragedia purtroppo rimasta viva per tanto tempo solo nel ricordo dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime. Un capitolo buio della nostra storia, per troppo tempo taciuto e negato, forse per il timore che la memoria di quegli eccidi suonasse impropriamente come una giustificazione dei crimini commessi dal regime fascista. Fu un grande Presidente della Repubblica, con un passato da partigiano nella resistenza al nazifascismo, Carlo Azeglio Ciampi, a sottolineare l'importanza del Giorno del ricordo. (cito testualmente) che quel giorno «testimonia la presa di coscienza dell'intera comunità nazionale. L'Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci anima il risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro. La responsabilità che avvertiamo nei confronti delle giovani generazioni ci impone ci impone di tramandare loro la consapevolezza di avvenimenti che costituiscono parte integrante della storia della nostra patria». Il dovere della memoria di quell'eccidio, come di tutte le altre sanguinose vicende dei totalitarismi, nasceva, per l'allora Capo dello Stato, dall'esigenza di difendere la civiltà europea, che è fatta di umanità, di rispetto per l'altro, di fede nella ragione, nel diritto e nella solidarietà, che la Seconda guerra mondiale ha rischiato di inghiottire. Il compito che noi abbiamo qui oggi è allora quello di nutrire la memoria della tragedia delle foibe, con iniziative rivolte alle nuove generazioni. noi voteremo a favore di questa proposta di legge, che, attraverso un concorso universitario, rivolto anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, prova ad istituire questo ricordo. Proviamo anche insieme a trovare le risorse per sostenere i viaggi delle scuole superiori, affinché di quell'eccidio rimanga la memoria, perché non debba più capitare. Questo anche perché riteniamo che, attraverso la scuola, l'università, il coinvolgimento delle giovani generazioni, possa esserci un vaccino potentissimo contro il rischio del contagio della violenza nazionalista, di qualunque segno ideologico e di qualunque colore. Abbiamo il dovere di ricordare, di non cancellare le tracce delle sofferenze patite dal popolo italiano, così come abbiamo il dovere di portare avanti un impegno per la verità, contro ogni reticenza ideologica o rimozione opportunistica. Da parte nostra, come parlamentari e rappresentanti del popolo, mi auguro che ci sia oggi la maturità che c'è stata vent'anni fa, da parte del Parlamento di allora, che istituì appunto il Giorno del ricordo. Mi auguro che ci sia una maturità analoga per fare un passo ulteriore il Parlamento agisca come allora, quando seppe convergere in modo quasi unanime su di una legge fondata sul rispetto e sull'amore per la verità e per i nostri connazionali. Allo stesso modo, io mi auguro che questo Parlamento approvi oggi a larghissima maggioranza questa proposta di legge, anche perché deve essere chiaro a tutti che i morti delle foibe non sono né di destra né di sinistra, ma sono cittadini vittime della storia di quegli anni e come tali vanno ricordati e rispettati. La storia italiana ed europea del secolo scorso è stata una storia di errori e di orrori, che occorre guardare in faccia senza equivoci e senza indulgenza. A qualificare, anzi a squalificare, il totalitarismo non è il colore rosso o nero, ma la natura di un regime politico senza rispetto per la vita, senza rispetto per la libertà e per la dignità umana. umana. Il ricordo dei morti delle foibe non cancella né redime le colpe mostruose di cui il regime fascista si macchiò nelle terre in cui migliaia di italiani furono torturati e assassinati dalle milizie titine e dove altre centinaia di migliaia furono costretti all'emigrazione forzata. Quella non fu una ritorsione per gli errori del regime fascista, perché gli innocenti ingoiati dalla profondità delle cavità carsiche nulla avevano a che vedere con il fascismo. Di cosa erano colpevoli? Di essere italiani. Anche certa propaganda, negli anni a seguire, non alleviò la sofferenza di quei 250.000 profughi, che in Italia cercavano solo accoglienza e comprensione. Ancora una volta, di cosa erano colpevoli? Erano solo italiani. E mi piace proprio quest'oggi ricordare l'impegno del presidente Giorgio Napolitano, che tanto ha fatto per restituire verità a quei tragici avvenimenti. Così come voglio ricordare, lo ha già fatto il collega De Cristofaro, l'impegno del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che proprio il 13 luglio del 2020 fu protagonista di una stretta di mano con il presidente sloveno Pahor alla foiba di Basovizza: un gesto semplice, ma pieno di significato. *(Applausi)*. In quell'occasione, il presidente la storia non si cancella, che possiamo coltivarla con rancore, oppure farne patrimonio comune nel ricordo. Noi sappiamo qual sia la strada da

Signor Presidente, come molti colleghi hanno ricordato, sono passati molti anni, circa venti, da quando è stato istituito il Giorno del ricordo, con una legge voluta dal Parlamento quasi all'unanimità: i voti contrari furono pochissimi e non sono un vanto per chi li espresse. Abbiamo prima ricordato il presidente Napolitano; con lui e altri Presidenti della Repubblica gli eventi della memoria hanno avuto importanza: spesso, anche negli ultimi anni, sono stati ospitati al Quirinale o in quest'Aula, dove abbiamo celebrato numerose volte il Giorno del ricordo con testimonianze varie. Non è ancora sufficiente, perché viviamo in un clima negazionista per certi versi. Ancora qualcuno rimbrotta chi vuole portare la memoria delle foibe

celebrando in questo modo il Giorno del ricordo - che servono a promuovere dei viaggi della memoria degli studenti nei luoghi delle foibe e dell'esodo. Si di cifre per la verità molto ridotte. Al Governo, negli anni, fatta la legge si può trovare non l'inganno, ma semmai la moltiplicazione delle risorse: dal museo

furono conservati, ora quelle masserizie, quei ricordi e testimonianze sono stati portati in un luogo più ampio, nel porto di Trieste, con un museo che è stato realizzato ma che può essere ancora ampliato, migliorato

della Foiba di Basovizza, dove avvenne il gesto simbolico del presidente della Repubblica Cossiga. Si dovettero attendere decenni per gesti simbolici in omaggio alle foibe e già questo fa capire quanto sia stata sofferta la riconquista di uno spazio nella memoria collettiva di una storia patria per troppo tempo negata.

conoscenza e ricordo; è finalizzato alle visite degli studenti, con programmi e gestione da parte del Ministero dell'istruzione, che ha già delle strutture e dei dirigenti che di questo si occupano. Abbiamo avuto una convergenza in Commissione e abbiamo dovuto limare qualche passaggio. Voglio anche dire che questo disegno di legge è un altro momento per una riscoperta di verità. Ci sono cose che vanno ancora accertate: nel 1946 a Vergarolla, sulla costa di quelle terre, ci fu una strage, la prima del Dopoguerra, e quindi non c'è stata soltanto quella di Portella della Ginestra, che giustamente viene ricordata; nel 1946 morirono su quella spiaggia tanti italiani. Poi si disse che erano esplosi dei materiali bellici che lì erano stati depositati. Noi riteniamo che anche il Parlamento debba fare accertamenti su una vicenda di questa natura ed auspichiamo che l'editoria sia più coraggiosa.

per dire loro quello che pensavo di quel negazionismo. Poi sul libro c'erano anche delle menzogne attribuite a me, che avrei detto che milioni di italiani erano stati uccisi nelle foibe. Non sono così ignorante

sede di cultura, dà alle stampe libri che contengono menzogne del genere. Poi hanno fatto un'altra stampa levando la menzogna. Noi siamo ancora in questo clima: non penso al volantino dei centri sociali negazionisti, o a quelli che impedivano a Giampaolo Pansa di presentare i libri sul triangolo della morte, che poi si estesero all'isola Calva e ad altre storie di tortura, di prigionia nella peraltro, prima si è parlato degli errori fatti nel passato da alcuni comunisti e sull'isola Calva venivano arrestati anche i comunisti italiani che evidentemente non erano considerati sufficientemente collaborazionisti, o che, dopo aver collaborato all'infoibamento dei loro connazionali, avevano avuto un conato di verità. Insomma, c'è ancora molto da dire e da scrivere, senza alcun revanscismo, senza voler seminare odio, ricordando tutte le tragedie del Novecento. È inutile dire disegno di legge non si contrappone ad alcun altro momento di ricordo, di memoria. Ci sono leggi dello Stato. L'Olocausto, nella sua dimensione, è una tragedia che non ha uguali per l'orrore che giustamente solleva e le scuole, il Parlamento e i mezzi di comunicazione ne parlano.

onorato di essere stato promotore di questo provvedimento che si è incrociato con le volontà di altri Gruppi del centrodestra, ma credo che la volontà del Parlamento sia unanime. Anche se

confrontato le opinioni di tutti e affermato il valore doveroso di una ricerca di memoria. Non aggiungo altro, non c'è bisogno di aggiungere affermazioni ulteriori. È un percorso importante e mi auguro che anche le norme sul negazionismo, che vengono giustamente applicate in alcuni casi, possano tutelare anche la memoria delle foibe e dell'esodo, per far sì che chi dovesse negarlo, che siano i libelli di Laterza o altri, incorra nei rigori non tanto della legge,

durante l'esilio statunitense nel 1947, lo stesso anno in cui esce «Se questo è un uomo» di Primo Levi. «Un sopravvissuto di Varsavia» è un oratorio per voce recitante della durata di soli sette minuti, che comincia con la seguente frase: «Non posso ricordare ogni cosa». Scriveva Iosif Brodskij in una prosa giustamente celebre: «La memoria tradisce chiunque, specialmente coloro che abbiamo conosciuto meglio. È un'alleata dell'oblio, un'alleata della morte, è una rete con cui si pesca poco e che non trattiene l'acqua. Non si può usarla per ricostruire qualcuno, neanche sulla carta». Se è vero che il passato è sempre lì e serve anche quando non hai più bisogno di ricordarlo, è altrettanto vero come la nostra epoca in particolare abbia bisogno di memoria, in specie se pensiamo alle giovani generazioni. Mi riferisco a quei giovanissimi considerati nativi digitali, ragazzi, cioè, che vivono in una connessione continua attraverso Internet, in un bisogno perenne di rincorrersi, sempre più esasperato dalla tecnologia che dà loro la possibilità di comunicare in ogni istante e in ogni luogo. Un primo dato positivo da segnalare è che, in modo diretto o indiretto, i tre disegni di legge riuniti in un testo unificato si rivolgano virtualmente proprio alle giovani generazioni, alle vittime designate, cioè, di quel progresso scorsoio di cui parlava il poeta Andrea Zanzotto. E chissà se proprio la maggiore consapevolezza non possa contribuire ad attenuare quel progressivo oscurarsi, cui abbiamo assistito e assistiamo, del futuro come promessa in un futuro come minaccia. In breve, pare lecito chiedersi se tanta demotivazione giovanile e forse anche tanta violenza non dipendano, pur dentro la difficile cornice in cui viviamo, da una scarsa conoscenza del passato che si proietta fino a rafforzarlo nel senso di buio in cui si concentra e sembra concludersi il futuro. Altro dato positivo, oltre al più generale lavoro di sintesi compiuto in Commissione, è stato che il Governo, d'accordo con il relatore e accogliendo un ordine del giorno dell'opposizione, rispetto a una tematica così importante quale la diffusione della conoscenza e della tragedia delle foibe, abbia acconsentito a sostenere ad ampio giro di compasso tutte le associazioni che hanno il merito di portare avanti pregevoli iniziative scientifiche, culturali e storiche. Si tratta di un passo importante per la memoria storica. Non posso non pensare al canto di Ulisse in «Se questo è un uomo», quando Primo Levi cerca di insegnare l'italiano a un compagno di prigionia recitando a memoria i versi del canto di Dante. A un certo punto Levi non ricorda, è disperato, perché comprende che dentro quella falla, in quei versi mandati a memoria che non riesce a mettere insieme, può racchiudersi il senso stesso dell'esistenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la letteratura, la testimonianza, la memoria, il documento storico, in particolare i frangenti storici possono assumere un significato importante per la difesa stessa della libertà interiore. Nel suo capolavoro «Un mondo a parte», lo scrittore polacco Gustaw Herling, riferendosi ai tentativi di fuga immaginati da alcuni prigionieri durante la Seconda guerra mondiale in un campo di lavoro sovietico, scriveva: «Prima della caduta di Parigi una donna alta con la testa e le spalle avvolti in uno scialle attraversava a quell'ora il piccolo tratto di strada visibile dalla finestra della cella, si fermava accanto a un lampione di fronte al muro della prigione ad accendere una sigaretta e spesso accadeva che alzasse il fiammifero acceso nell'aria come una torcia e lo tenesse un attimo in quella posizione incomprensibile. Decidemmo che quello era un segno di speranza». Anche quello delle foibe fu un mondo a parte, una fra le pagine più buie e forse in parte ancora da conoscere a pieno, decifrare, ricordare, sicuramente diffondere nei libri di storia e collocare tra le pieghe più sottili e nascoste del Secolo breve del passato prossimo novecentesco e non può essere concentrato solo nella opacità di una diapositiva sfocata o nella volatilità del *wallet* di un cellulare. In ogni momento della nostra vita noi possiamo comunque decidere che una pagina, un verso, un racconto, un'immagine, un documento storico, una testimonianza riescano in fondo a far luce, rimangano insomma come quel fiammifero acceso nell'aria, si trasformino e divengano per noi motivo di riflessione, auspicio di verità e segno di speranza. Per questi motivi, signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole a questo provvedimento.

Signor Presidente, colleghi, voglio esprimere subito la grande soddisfazione per l'approdo di questo disegno di legge in Aula. La 7a Commissione ne ha avviato l'esame appena insediata e ha approvato il testo frutto di un lavoro ben orchestrato del relatore, senatore Paganella, che ringrazio perché è riuscito a cucire dei provvedimenti analoghi, in parte difformi per le sensazioni, ma che andavano in un'unica direzione, dei senatori Romeo, Menia e Gasparri. Abbiamo avuto la pazienza di attendere i provvedimenti, che si intrecciassero, che venissero in Commissione, che fossero elaborati e grazie all'intera Commissione e alle forze politiche tutte si è arrivati a un testo congiunto, un testo validato da tutti i i partiti politici. Ritengo fosse doveroso prevedere attività capaci di rendere sempre vivo il ricordo di questa tragedia che ha vissuto il nostro Paese. Ringrazio chiaramente anche

inghiottitoi naturali, molto diffusi nelle zone carsiche. La cavità si restringe, scendendo in profondità, per poi chiudersi e riallacciarsi in un bacino: una forma che rende difficili la risalita e i soccorsi. Gli eccidi delle foibe, commessi dai partigiani jugoslavi, vedevano le vittime spesso gettate vive in quelle cavità. La storiografia distingue due ondate di La prima risale al settembre del 1943, quando il fascismo cade e l'Italia firma l'armistizio con i tedeschi che occupano in un primo momento solo i centri ritenuti d'importanza strategica, come Trieste, Pola e Fiume;

rappresentative della comunità italiana come avvocati e levatrici. Dal furore iniziale, la violenza divenne più programmata al fine di ripulire il territorio per eliminare ogni ostacolo alle affermazioni di un nuovo corso politico. Non mancarono i linciaggi così come le violenze sessuali. La seconda ondata di violenze di massa iniziò poi a maggio del 1945, nel momento in cui le truppe jugoslave entrarono nella Venezia Giulia, perseguendo lo stesso obiettivo: eliminare chiunque si potesse opporre all'egemonia di Tito, tanto che non mancarono numerosissime vittime anche tra croati e sloveni non in linea con i comunisti. Il 10 febbraio è stato eletto, con legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Giorno del ricordo, perché proprio in questa data del 1947 furono firmati i Trattati di pace a Parigi con i quali si assegnavano l'Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli-Venezia Giulia alla Jugoslavia. I territori in questione erano stati assegnati all'Italia con il Patto di Londra, mentre la Dalmazia venne annessa a seguito dell'invasione nazista in Jugoslavia. Con il ritorno di questi territori alla Jugoslavia ebbe inizio una rappresaglia feroce che colpì molti concittadini italiani innocenti, ritenuti implicitamente colpevoli di aver vissuto sotto il regime fascista, fino a configurare quella che oggi gli storici descrivono come una vera e propria pulizia etnica con prigionia, campi di lavoro forzati e morte nelle foibe, che coinvolsero tra le 4.000 e le 5.000 persone. Molti riuscirono a fuggire: un esodo di massa che coinvolse tra le 250.000 e le 350.000 persone tra il 1945 e il 1956, in meno di undici anni. Non vi è dubbio che i motivi di tanta violenza vanno ricercati non solo in un fatto scatenante, ma anche in una lunga scia di accadimenti che non hanno fatto altro che creare tutte quelle contrapposizioni antiche, nazionalistiche e politico-ideologiche che da sempre sono foriere di sangue e morte. Che ogni guerra porti dietro di sé uno strascico fatto di rese dei conti è la storia a dirlo: solo che in questo caso l'obiettivo era l'annichilimento del dissenso di tutti coloro che si sarebbero potuti frapporre alla presa del potere dei comunisti. Per questo, accanto al Giorno della memoria, dedicato alle vittime dell'Olocausto, è importante diffondere e valorizzare il Giorno del ricordo,

affinché nessuna sofferenza e nessuna brutalità siano più negate e simili atrocità non abbiano a ripetersi. La Lega con tale proposta, a firma del capogruppo Romeo, intendeva raggiungere questo obiettivo, istituendo un concorso annuale per la realizzazione di una installazione permanente, in ricordo del dramma delle foibe, da esporre per la durata di un anno in uno dei tanti capoluoghi di Regione italiani. L'arte è un potente strumento di pace, può parlare alle coscienze più di mille parole e contribuire a non perdere il ricordo di eventi storici anche terribili come questi e a sensibilizzare le coscienze affinché non si ripetano più. La memoria parla al cuore per comprendere in profondità quanto male hanno procurato le ideologie di parte, le dittature, la guerra e tutto l'odio che ne è seguito: questo obiettivo si raggiunge anche attraverso l'arte e la bellezza, armi potenti, anzi potentissime, che rendono sterile l'odio. *(Applausi)*. Sono contento che a questa previsione si siano aggiunte quella dei colleghi Gasparri e Menia, che prevedono rispettivamente la creazione di un fondo di un milione di euro per permettere l'organizzazione di viaggi del ricordo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e uno stanziamento di fondi in favore delle associazioni degli esuli, che ancora oggi rappresentano la memoria di quei tragici eventi e contribuiscono in maniera importante a tramandarla. Credo che questo disegno di legge porti un contributo importante al nostro Paese, in cui le ferite lasciate dalla guerra non si sono ancora rimarginate e dove un vero e proprio percorso di pacificazione non è stato ancora compiuto; dove ancora vivono le contrapposizioni alimentate dall'incapacità di superare le appartenenze ideologiche. Per questo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, nel 2004 è stato istituito il Giorno del ricordo con una legge che ha voluto ricordare una delle grandi tragedie di quel martoriato lembo di terra chiamato un tempo confine orientale, dove sono nata e dove vivo; una legge che ha voluto anche porre le basi per una riconciliazione nazionale e credo che chiunque venga chiamato a prendere la parola in tal senso debba tenerne conto. Non onora le vittime chi si serve di questa tragedia per fare propaganda politica, o peggio ancora chi, pur ricoprendo importanti ruoli istituzionali, pensa a scattarsi dei *selfie* durante la cerimonia del Giorno del ricordo al monumento della foiba di Basovizza, com'è successo. *(Applausi)*. Strumentalizzare questa tragedia è un errore, un peccato gravissimo che contraddice lo spirito stesso della legge, votata peraltro allora in Parlamento quasi all'unanimità. Questi decenni hanno segnato un cambio di passo in quel percorso di amicizia e collaborazione tra due comunità, due Nazioni, due Paesi confinanti che tutti dobbiamo impegnarci a consolidare. Nella giornata del 13 luglio del 2020, i presidenti delle Repubbliche di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, hanno posto Trieste al centro del mondo, tenendosi per mano in due luoghi simbolo del Novecento giuliano per guardare al futuro. È stata quella delle nostre terre un'epopea tragica e gloriosa nel contempo, in cui la scelta di stare dalla parte dei giusti e di lottare per la libertà, una libertà che non è appannaggio di alcuni soltanto, ma il bene supremo, non può essere in alcun modo confusa, rivista o messa in dubbio, nonostante i drammatici eventi di Arbe o Gonars, due campi del duce; nonostante gli orrendi crimini commessi durante l'occupazione dei fascisti di parte della Jugoslavia; nonostante la risiera di San Sabba e nonostante la tragedia dei morti delle foibe e dell'esodo. Lo ricordava il presidente della Repubblica Mattarella, che ha lottato per la libertà ed è un esempio per tutti: chi vorrebbe scambiare i ruoli tra le vittime innocenti e i nazifascisti, chi vuole tentare un revisionismo storico, commette un peccato mortale nei confronti non nostri, ma di milioni di morti. Non credo nella memoria condivisa: credo invece nel rispetto delle singole memorie. Ciascuno di noi ha il diritto di piangere i propri morti, perché ogni morte è assenza e dietro a ogni morte ci sono madri e padri, sorelle e fratelli, mogli e mariti, figli che resteranno segnati e in tal senso per sempre - da quell'assenza. *(Applausi)*. La memoria storica rappresenta il nostro futuro. Il Giorno del ricordo non può dunque diventare monopolio della destra o dei suoi esponenti, soprattutto in luoghi significativi che ne determinano la sacralità. Per noi questo è motivo di profondo rammarico, perché dobbiamo rispetto alle vittime e agli esuli. Tragedie così grandi non si utilizzano al fine di ottenere un consenso per se stessi o per la propria parte politica. Nella memoria dolorosa si ha il dovere di entrare con il passo rispettoso, senza forzature e senza l'intendimento di voler imprimere il proprio marchio politico alla tragedia di migliaia di persone, che passa in seconda linea o, peggio, viene dimenticata o strumentalizzata. È importante non dimenticare: non dimenticare chi ha dovuto lasciare tutto e cercare di ricostruire una vita altrove; non dimenticare i morti per mano dell'ideologia, non per odio etnico. Io nasco da una famiglia antifascista che ha sofferto come tutta la mia comunità per le violenze e i soprusi durante il quarto di secolo fascista e nazista e che ha pagato cara la propria appartenenza nazionale e quindi il proprio anelito alla libertà. Ho frequentato le scuole con lingua e insegnamento sloveno, istituzioni e associazioni, ma non ho mai sentito una sola parola di odio o di indifferenza nei confronti di chi ha sofferto le nostre pene, di chi ha dovuto, come oltre 100.000 sloveni durante il periodo fascista, abbandonare la propria propria casa e la propria terra. Il diritto di Patria è una cosa seria e va rispettato e onorato. *(Applausi)*. È importante per le più alte istituzioni parlamentari, la Camera e il Senato della Repubblica, non abbandonare al monopolio di una parte politica un discorso storico che ha permesso una legge votata anche dal centrosinistra nel 2004. La strumentalizzazione fatta da alcuni esponenti della destra nei luoghi sacri, come sono le foibe, consiste anche nell'enfatizzare oltre misura la componente nazionalistica che emerge dalla contrapposizione italiani, slavi e, quindi, comunisti e anti-italiani. Gli eccidi del secondo Dopoguerra hanno toccato tutti in Italia, in Slovenia e in Europa. Non dimentichiamocelo e non dobbiamo disinteressarci di questo. La strumentalizzazione della tragedia post-bellica, quello che veniva chiamato confine orientale è segnata molto dall'offensiva spregiudicatezza di alcuni. Il ministro Salvini a Trieste è riuscito a parlare di bambini infoibati, un falso storico totale. Non si può né si deve colpevolizzare gli infoibati e gli esuli per quanto successo prima, per i crimini del fascismo perpetrati per un quarto di secolo. Si deve invece partire dal presupposto insindacabile che chi è morto o è scappato è una vittima delle dittature che si sono susseguite e hanno definito la storia della mia terra amata e offesa più e più volte. La Storia con la s maiuscola è fatta di tante storie che segnano i destini delle persone; di questo dobbiamo avere rispetto e ci fosse stata una sola vittima innocente, prima, durante o dopo la guerra, sarebbe stata troppo. Le memorie sono diverse, ma ora noi tutti, cittadini europei di quel confine orientale di un tempo, abbiamo costruito un cammino di pace, di amicizia, di libertà e di rispetto. Chi vorrebbe inficiare tutto questo non fa bene al proprio Paese. Sono grata al destino di aver vissuto questo momento storico in cui non debbo più avere timore di parlare nella mia lingua madre per certe strade di Trieste, per non farmi prendere a schiaffi, sputi o insulti, come mi è successo a diciassette anni, e ricordo bene per mano di chi. Ebbe a dire Luciano Violante che ricordare vuol dire capire, anche se capire non vuol dire condividere. Oggi ci accingiamo ad approvare un disegno di legge importante, e il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. Credo che per approfondire certi aspetti di queste vicende sarebbe bene riprendere in mano il testo della relazione della commissione mista storico culturale italo-slovena, i cui esponenti di destra e di sinistra hanno lavorato dal 1993 al 2001: ripartire, approfondire, riconoscere, ristudiare. In questa ottica, ci risulta difficile comprendere l'atteggiamento di una parte della maggioranza, contrario all'approvazione di alcuni emendamenti che abbiamo proposto per definire un nuovo finanziamento anche ad associazioni (tra le quali vorrei citare il Circolo Istria) che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'alto Adriatico. Ci sono stati e ci sono ancora esuli istriani e dalmati, che hanno condiviso la necessità di un approfondimento, ma non hanno aderito all'idea di strumentalizzare questo discorso e soprattutto questa tragedia. Sono forse questi, considerati di sinistra (quasi fosse una colpa), meno esuli di altri? Vorrei ricordarne due tra tutti, compianti sindaci del mio Comune, Giorgio Depangher e Marino Vocci, che hanno cominciato un dialogo splendido e costruito amicizie amicizie e collaborazioni, in un clima di rispetto reciproco tra tutti noi. E mi sia permesso ricordare - come è già stato fatto - con un commosso pensiero Norma Cossetto, di cui il prossimo 5 ottobre ricorderemo l'ottantesimo anniversario della tragica fine. Voglio concludere con le parole di un grande premio Nobel per la pace, Nelson Mandela: «Le menti che cercano vendetta distruggono gli Stati, mentre quelle che cercano la riconciliazione costruiscono le Nazioni. Uscendo dalla porta del carcere verso la mia libertà, sapevo che, se non mi fossi lasciato alle spalle tutta la rabbia, l'odio e il risentimento, sarei ancora prigioniero». Signor Presidente, colleghi, vi dirò che questa dichiarazione di voto per me non non è certo banale come altre, non è l'ultimo atto scontato del rito della liturgia parlamentare. Oggi per me è molto di più, perché perché questa è una cosa che a me sta nel cuore. Come ho avuto modo di dirvi molte volte, io sono figlio di quell'esilio istriano, orgoglioso figlio di quell'esilio istriano, che so a chi devo. a chi devo. Per me questo è un fatto che anche intimamente muove il cuore e la coscienza. E allora voglio dirvi che questa per me è un'altra tappa comunque di vittoria di una vecchia battaglia di giustizia contro la congiura del silenzio, contro il negazionismo, contro il giustificazionismo, che anche oggi ho sentito aleggiare più e più volte. Non mi voglio quindi limitare - come è ovvio -

che poi dice tante cose. Ma in particolare - a mio modo di vedere - segna il passo ed ha più significato, perché

Parlando di questi luoghi, non posso che cominciare da Basovizza. Per chi di voi non lo sapesse, Basovizza, secondo la definizione di quello che fu un grande vescovo di Trieste (anzi, era vescovo di Trieste e Capodistria, perché allora le diocesi erano unite), monsignor Santin, è un calvario con il vertice sprofondato nelle viscere della terra. E nelle viscere della terra, lì, ci sono 500 metri cubi di infoibati, che vuol dire 2.000 vite finite là sotto. Era il maggio del 1945; quella foiba fu chiusa nel 1959. Trieste era ritornata all'Italia cinque anni prima. Era passato il Governo militare alleato e in tutti quegli anni era la discarica degli abitanti di Basovizza. Nel 1970 fu posta una nicchia, all'interno della quale c'erano i 4.361 nomi di infoibati e deportati di Trieste e dalla Venezia Giulia, raccolti dal sindaco della seconda redenzione Gianni Bartoli. Il 3 novembre del 1991 per la prima volta un Presidente della Repubblica italiana si degnò di venire a Basovizza: era Francesco Cossiga. Erano passati quasi cinquanta anni. *(Applausi)*.

che ho vissuto in Parlamento. Ottanta anni dopo - pensate a quanto tempo maledettamente è passato - porteremo i ragazzi a vedere Basovizza. Fino ad oggi ci venivano, ma ci venivano volontariamente o con quei professori che, con l'ostilità di altri professori e del corpo docente, li portavano a vedere Basovizza. Oggi lo farà, finalmente, lo Stato. Quanto tempo! Quanta pazienza! Quanta perseveranza! Catone il vecchio, *Cato* *censor*, ci insegnava che la pazienza è la più grande di tutte le virtù. La tradizione cristiana ci ha trasmesso che è la virtù dei forti e, anzi, sant'Agostino diceva che ad essa si sommava il dono della perseveranza. Noi abbiamo avuto pazienza e perseveranza.

La canta Dante nel canto IX dell'Inferno: «Sì com'a Pola, presso del Carnaro ch'Italia chiude e suoi termini bagna». A Pola sorge una grande arena, che è nata prima del Colosseo, anche se non lo sa quasi nessuno. In quel febbraio del 1947, 32.000 polesani su 34.000 abitanti se andarono per sempre. Partirono col piroscafo Toscana. Sul Toscana stava il vescovo Radossi, che celebrava la messa sul ponte, quando partivano e salutavano con la bandiera Pola, che non avrebbero rivisto mai più. E cantavano

se la stampa, che sa consacrare colonne di prima pagina ad un processo, non sa occuparsi delle vostre lacrime. Lasciate fare al tempo, che è sempre stato medico e maestro impareggiabile.

quando si parla della storia di un popolo che è stato sradicato, che ha subìto una grande ingiustizia, la pulizia etnica e un grande esodo. Il tempo uccide la memoria e la storia dei popoli. Ne decreta la scomparsa, tradisce il ricordo. Il tempo cancella tutto. Ecco perché forse questa è la maledizione del tempo. Parlando di questi luoghi, essi diventano monumenti attraverso il passare del tempo. Monumento deriva dal latino, dal verbo *monere*, che vuol dire ammonire, che vuol dire ricordare. Parliamo di luoghi che diventano monumenti e poi parliamo di luoghi che sono bruciati ormai dal tempo, perché non sono e non saranno mai più quello che erano.

il campo profughi di Padriciano. Mi ricordo quando andai lassù con una donna, si chiamava Fiore, che mi raccontò di sua sorella Marinella, che nell'inverno del 1956 morì di freddo. Non aveva neanche un anno. La mamma la portò al medico del campo, era diventata tutta blu, e il medico le disse: signora, sua figlia è morta di freddo. Dietro quei campi profughi però si stava nel filo spinato, nelle baracche, e in quegli stanzoni in cui le famiglie venivano divise da coperte che venivano attaccate in alto, ai soffitti, attraverso il filo di ferro. Quei campi profughi sono stati

medaglia d'oro al valor civile conferita dal presidente Ciampi il 9 dicembre 2005. Accompagnai sua sorella - quanto le volevo bene - che mi raccontò tutto di quella storia. Altro che certe interpretazione dei fatti e il loro utilizzo; quante ve ne potrei raccontare. Sapete cosa dice la medaglia d'oro? Così recita: «Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Villa Surani».

Parliamo di Ernesta e di Zulema Adam, moglie e figlia di Angelo Adam, ebreo di Fiume, socialista, ma italiano? Era tornato da Dachau, dov'era sopravvissuto (tatuato

con il suo cagnetto bianco». Parliamo di Giuseppe Librio, che si arrampica a Fiume su piazza Dante per mettere il tricolore e gli sparano nella tempia? Fatemi ricordare Nidia Cernecca, a cui volevo tanto bene e che, con un coraggio da leone, andò a inseguire Ivan Motika, il boia di Pisino, che aveva portato a morte centinaia e che fece rapire, ad esempio, Don Angelo Tarticchio. Vogliamo parlare dei trentasette preti ammazzati? Don Angelo Tarticchio fu trovato in una cava di bauxite, infoibato, nudo, con i genitali in bocca e una corona di spine calata sulla testa. Vogliamo parlare del beato Francesco Bonifacio, di Villa Gardossi, di Buie d'Istria, che è la città di mia mamma? È colui che scrive che chi non ha il coraggio di morire per la sua fede non è degno di professarla. Queste sarebbero libere interpretazioni della storia?

Adesso vi leggo un'ultima cosa, davvero l'ultima, ma ve la voglio leggere. È un'altra storia di un eroe, una storia che viene da Cherso: bellissima Cherso, veneziana, con i suoi leoni di San Marco, nel Quarnaro, isole Absirtidi, perché là corre il mito di Medea e Giasone e del vello d'oro. È la storia di un giovane eroe che si chiamava Stefano Petris, un maestro di lettere costituì una sua compagnia per difendere Cherso. Si chiamavano quelli della tramontana; si ribellò ai tedeschi e combatté contro di loro che volevano ammainare il Tricolore d'Italia. Là morì il primo dei suoi, che si chiamava Giovanni Negovetti, a diciott'anni, contro i tedeschi. Poi difese Cherso jugoslavi, dai partigiani di Tito; era il 20 aprile del 1945, quando ormai la città era perduta, tutto bruciava e le strade erano fiumi di sangue ed era rimasto un pugno di uomini e ferito per la terza volta si consegnò prigioniero. Verrà fucilato a guerra finita, poco prima del Natale 1945. La notte prima di essere ucciso, scriverà le seguenti parole a sua moglie sul retro dell'ultimo foglio sgualcito de «L'imitazione di Cristo», che teneva sempre con sé: «Non piangere per me. Non mi sono mai sentito così forte come in questa notte di attesa, che è l'ultima della mia vita. Tu sai che io muoio per l'Italia. Siamo migliaia di italiani gettati nelle foibe, trucidati e massacrati, deportati in Croazia, falciati giornalmente dall'odio, dalla fame e dalle malattie, sgozzati iniquamente. iniquamente. Aprano gli occhi gli italiani, puntino i loro sguardi verso questa martoriata terra istriana che è e sarà italiana. Se il Tricolore d'Italia tornerà, come spero, a sventolare anche sulla mia Cherso, bacialo per me, assieme ai miei figli. Domani mi uccideranno, ma non uccideranno il mio spirito né la mia fede. Andrò alla morte serenamente e come il mio ultimo pensiero sarà rivolto a Dio che mi accoglierà e a voi che lascio, così il mio grido fortissimo, più forte delle raffiche dei mitra, sarà: viva l'Italia!».

di amore e di dolore, di morte e di vita, e a tramandare queste lettere e a ricordare questi eroi, donne e uomini, martiri e santi, noi avremo vinto la maledizione del tempo.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

come abbiamo appena sentito, la memoria è radice di una comunità e fare memoria è la condizione perché la storia umana e i suoi errori non si ripropongano e perché si possano invece rinsaldare i legami e i valori di una comunità. Oggi ricordiamo i dieci anni da un episodio drammatico, in cui persero la vita 368 persone a Lampedusa

Pensiamo che quei corpi, signor Presidente, colleghi, ci dicano ancora una verità e cioè che il Mediterraneo è stato, è e deve continuare a essere una culla di civiltà e, come ha detto il Papa, culla significa vita, pertanto non è tollerabile che diventi una tomba e nemmeno è tollerabile che il Mediterraneo diventi luogo di conflitto e di scontro di civiltà. Il Mediterraneo è

ricordo che già nel 2013, quando ero Ministro del Governo Letta, facemmo partire l'operazione Mare nostrum; poi nel 2015 ci fu un'altra tragedia terribile, con oltre 700 persone morte, e volemmo recuperare la nave sui fondali del Mediterraneo proprio perché non si perdessero la memoria e il ricordo di quella tragedia. Questa memoria ci dice anche che l'Europa è chiamata a fare un salto di qualità, di qualità, nella sua umanità, nei suoi valori fondanti e nella sua azione per un'immigrazione che non è un fenomeno congiunturale, ma strutturale. Quelle persone morte ci chiedono di fare un salto politico e di togliere dalla polemica politica la strumentalizzazione delle speranze, delle ansie e dei desideri di tante migliaia di persone che cercano un futuro migliore per sé e per le loro famiglie. Non c'è nulla da temere da queste speranze, l'Europa non deve temere nulla da persone - donne, bambini e adulti - che vogliono venire qui per lavorare e per costruire un futuro migliore, come hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni.

che non sia né di destra, né di sinistra, ma che semplicemente possa aiutare questo Paese, finalmente, ad affrontare quello dell'immigrazione come un problema vero, sostanziale sostanziale e strutturale del nostro Paese, con misure serie che favoriscano l'immigrazione legale, che diano cioè concretezza e sostanza ai sogni di tante persone, che prima di tutto, come ci ricordano quei corpi,

10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione